Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

questo provvedimento, collegato alla finanziaria, ritorna qui in Senato in quarta lettura. Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati il 1° luglio hanno riguardato 13 articoli sui 64 del provvedimento, ed alcune di esse sono di contenuto veramente marginale. Con il suo permesso, signor Presidente, lascerei la relazione agli atti, perché i colleghi conoscono bene la problematica.

1195-B ritenendo che il provvedimento, che ricordiamo è un collegato alla finanziaria, nel corso dell'esame parlamentare al Senato e alla Camera (il collega Paravia prima ricordava che siamo in quarta lettura)

- alla norma contenuta nell'articolo 64, recante disposizioni in materia di farmaci, come pure ad altre disposizioni, contenute negli articoli 58 e seguenti, in materia di trasporto ferroviario. Risultano poi anche presenti nel provvedimento alcune norme che recano delle vere e proprie deleghe in bianco al Governo, prive di qualsiasi oggetto esattamente determinato, e ciò in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che, lo ricordo, recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». presente, come ho già detto all'inizio del mio intervento nell'illustrazione della questione pregiudiziale, che la risoluzione di approvazione del DPEF 2009-2013

intimamente funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria e, in quest'ottica, oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto di tali provvedimenti. Si indicano, infatti, come collegati i disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria ed i Regolamenti parlamentari di Camera e Senato dettano una specifica disciplina dello *status* procedimentale dei provvedimenti collegati. In particolare, viene precisato che tali provvedimenti devono essere indicati nel DPEF, così come approvato dalla risoluzione parlamentare. Pare dunque al Gruppo dell'Italia dei Valori che questo e tanti altri motivi giustifichino la questione pregiudiziale che è stata posta. Riteniamo infatti palese che, nel caso in esame, abbiamo di fronte un provvedimento collegato che va ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF. Da ultimo, ma non per importanza, esso non è dotato di adeguata copertura finanziaria, come dimostrato anche dalla Nota tecnica inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati, in data 5 5 giugno 2009. Vorrei leggervi il dispositivo della nota tecnica inviata dal Ministero: «nel disegno di legge (...), oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico-finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione». Il dispositivo che vi ho appena letto non è stato scritto del Gruppo Italia dei Valori, ma - lo ripeto - è una nota tecnica inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Camera dei deputati il 5 giugno 2009. Per i suddetti motivi, chiediamo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, non si proceda all'esame dell'atto Senato 1195-B.

le Regioni e gli enti locali nei procedimenti autorizzativi determineranno una lesione di competenze costituzionamente definite. Segnalo altresì che tali previsioni determineranno l'accentuarsi di un conflitto Stato‑Regioni, che sicuramente non gioverà a garantire speditezza e velocità nell'assunzione delle necessarie decisioni per il rilancio economico del

privo di risorse finanziarie e molte delle norme non risultano coperte o enunciano meccanismi applicativi che determineranno

Signor Presidente, interverrò brevemente perché invece penso che questo provvedimento debba proseguire il proprio corso presso il Senato e diventare finalmente legge. Si tratta infatti di norme importanti per il nostro Paese: il rilancio della nostra

inclusi quelli citati nella questione pregiudiziale, vanno precisamente in questa direzione.

per gli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. È particolarmente necessario riunire in un solo testo tutti i numerosi adempimenti, che si spera diventino sempre meno anche grazie

Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, gli occhi del mondo sono rivolti oggi all'Italia dove si svolge il Vertice dei grandi Paesi della terra che, tra le sue priorità, ha proprio la crisi e lo sviluppo. Nel contesto internazionale gli effetti della grave congiuntura che stiamo attraversando consentono però di rivalutare i presupposti su cui si basa la crescita italiana, inferiore nel *trend* rispetto ad altre Nazioni, ma più solida ed equilibrata. Questo è il frutto della propensione al risparmio delle famiglie italiane e della solidità del nostro settore manifatturiero. Le misure adottate dal Governo a favore dello sviluppo con il disegno di legge n. 1195-B al nostro esame sono, quindi, quanto mai idonee a sostenere la nostra economia perché rivolte proprio a famiglie ed imprese attraverso strumenti che rendono più innovativo, competitivo ed equo il nostro contesto socio‑economico. Riporto solo alcuni esempi che possono però dare la giusta misura della validità del provvedimento in questione. Il primo articolo del disegno di legge riguarda i distretti produttivi e le relative imprese che favoriscono aggregazione e accordi. Il testo del provvedimento consente la semplificazione dei processi di aggregazione e li rende convenienti per le imprese stesse. A favore di imprese e cittadini sono poi le misure adottate in materia energetica. Al riguardo il disegno di legge definisce una visione di interesse nazionale, delegando al Governo una funzione d'indirizzo degli interessi statali nel rispetto dei principi del titolo V della Costituzione: libertà di azione per le Regioni coerentemente con le esigenze del Paese e con le strategie di sviluppo condivise. In questo quadro s'inserisce il tema del nucleare, un cambio epocale non solo dal punto di vista economico ma anche con riferimento allo stile di vita degli italiani, perché strettamente collegato anche a processi di innovazione di prodotto orientati al risparmio energetico e alla sicurezza e, allo stesso tempo, alla ripresa e allo sviluppo.

Il risparmio giornaliero di cui che gli italiani stanno usufruendo in questo periodo ne è una dimostrazione. Ci sono poi una serie di misure attinenti ai distributori stradali di GPL che migliorano e rendono più sicuro il sistema distributivo e, allo stesso tempo, permettono ad un maggior numero di cittadini di usufruire dei vantaggi di questo sistema. Di rilievo anche l'estensione del contributo statale per l'installazione dell'impianto GPL ad ulteriori categorie di vetture, che si rivelerà di sicuro vantaggio. ma solo per dovere di sintesi, l'internazionalizzazione - di cui anche il collega Malan ha precedentemente parlato - con la delega al Governo, prevista nell'articolo 3, relativa alla raccolta e al coordinamento di tutte le disposizioni legislative in materia. Quanto previsto in questo provvedimento non farà altro che incentivare e rafforzare la naturale tendenza delle nostre imprese ad affacciarsi sui mercati. Ovviamente, non meno importanti sono tutti gli altri punti del provvedimento, che ha il pregio di snellire e razionalizzare l'impianto delle regole che sta alla base del nostro sistema economico e, allo stesso tempo, di agevolare le condizioni di vita di milioni di cittadini.

nonostante il Governo abbia avuto una seconda possibilità di sanare i rilievi denunciati dai funzionari della nostra amministrazione pubblica, nulla è stato fatto per risolvere questa contraddizione.

che attraverso tale inciso normativo la disposizione si rende suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, posto che estende la possibilità di accedere a forme incentivanti anche a quelle imprese che di fatto non hanno i requisiti per beneficiarvi". Questa parte del testo, nonostante tale invito, non è stata modificata in seconda lettura, è rimasta identica in terza lettura e ora che siamo alla quarta lettura, in ossequio al principio della doppia conforme, non si può più modificare. un'altra disposizione rimasta immutata nel testo del provvedimento, si legge: "La disposizione è altresì onerosa," - è sempre il Ministero dell'economia e delle finanze che scrive "con conseguenti profili di illegittimità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estensione delle misure finanziarie ed in materia di ricerca e sviluppo anche alle reti di imprese, senza prevedere adeguata copertura finanziaria". Più esplicitamente di così non si potrebbe In riferimento, infine, e cito soltanto l'ultimo caso, all'articolo 5, volto ad introdurre una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, la nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze addirittura si spinge a chiedere la soppressione della norma ex articolo 81 della Costituzione. Ci sono altri esempi di caratura minore, ma quelli più importanti sono questi. Se ne ricava che il Governo e la maggioranza ci chiedono di licenziare un provvedimento privo di copertura finanziaria, cioè si fanno le cose senza i soldi. Ovviamente il Governo e la maggioranza non possono stampare carta moneta, però invitano la società che si riferisce a queste leggi a ragionare in termini di moneta immaginaria. A questo siamo costretti. Noi siamo invitati dal Governo e dalla maggioranza a vivere in un mondo virtuale dove la moneta è immaginaria. Il Governo e la maggioranza ne traggano le conseguenze.

poiché l'argomento ci è noto e le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati non sono particolarmente significative ho pensato, per snellire l'approvazione

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che nel corso del suo esame, dall'agosto 2008, ha subito notevoli modificazioni, sino ad arrivare al testo attualmente in discussione. Un testo che contiene numerose disposizioni tra loro non collegate in un quadro normativo di complicata lettura, notevolmente disarticolato e in alcune parti di difficile applicazione. Il tutto per effetto di un modo di procedere del Governo, senza un preciso filo conduttore, ma in ragione di singole necessità e senza una visione di insieme, che sarebbe necessaria in provvedimenti di questa portata e rilievo: basti pensare alle norme sulla *class action,* sul trasporto ferroviario o sulle assicurazioni. Troppe e numerose sono anche le deleghe conferite al Governo, secondo un disegno volto probabilmente sempre più a svuotare il Parlamento delle sue funzioni con riguardo a scelte legislative che vanno ad incidere pesantemente sulla vita dei cittadini e sui poteri delle autonomie locali. Penso, in particolar modo, alla delega sul nucleare, che prevede l'adozione di decreti legislativi *ad hoc* per indicare i criteri di localizzazione sul territorio italiano degli impianti di produzione dell'energia nucleare e degli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. È questo uno solo dei tanti punti critici di un intervento complessivo che si pone l'obiettivo di rivedere le politiche energetiche nazionali attraverso la reintroduzione del nucleare, senza affrontare però il tema più ampio, legato all'approvvigionamento delle risorse energetiche e allo sviluppo di infrastrutture in tal senso. Il nostro Paese, che dipende per la gran parte da fonti energetiche di provenienza estera, avrebbe invece bisogno di investire sullo sviluppo di fonti alternative di produzione per migliorare il *mix* delle fonti nel breve periodo, senza attendere i tempi lunghi della realizzazione e dell'entrata in funzione delle centrali nucleari. Per questo le nostre proposte, presentate in sede di seconda lettura del provvedimento, si sono rivolte nel senso di incrementare e migliorare il *mix* delle fonti e di dare impulso al risparmio energetico, alla cogenerazione e alla generazione di piccola taglia. A tal proposito, vorrei anche sottolineare che il testo in esame contiene norme che, al contrario, aggravano i costi di autoproduzione dell'energia elettrica e disincentivano la cogenerazione, soprattutto di piccola taglia, anche in contrasto con le normative europee. Mi riferisco, in particolare, a quanto contenuto nell'articolo 33 in materia di reti interne di utenza, per le quali abbiamo presentato un apposito ordine del giorno. Se volessimo poi soffermarci sulle potenzialità di sviluppo e crescita economica che provengono dal settore energetico, potremmo asserire che la strategia vincente sta nel valorizzare gli investimenti in ricerca e innovazione in questi settori per sviluppare tecnologie nostre, che fanno da capofila di filiere nazionali e vengono anche esportate. Questo vale per le fonti alternative, tra cui le rinnovabili, e dovrebbe valere anche per il nucleare. Fare investimenti sul nucleare senza accompagnarli con un adeguato piano industriale per potenziare tutta la filiera nazionale, dalla ricerca alla progettazione, per arrivare alla realizzazione degli impianti, significherebbe mancare di una visione strategica d'insieme, la cui carenza non è compensata dalla supposta riduzione del costo dell'energia prodotta dal nucleare. Da come si sta muovendo questo Governo, invece, sembrerebbe che le uniche beneficiarie dell'opzione nucleare in termini industriali saranno le imprese francesi. Rispetto a quanto contenuto in questo disegno di legge ben altre dovrebbero essere le misure da adottare per rendere effettiva la concorrenza nei mercati dell'energia, con particolare riferimento al mercato del gas naturale, dove ancora persiste una situazione di monopolio di fatto. Le nostre proposte in tal senso sono state chiare nel corso dell'esame del provvedimento, sempre concentrate nell'ottica di favorire l'apertura del mercato, anche, per esempio, per ciò che concerne i tetti *antitrust,* di cui abbiamo chiesto la proroga. Inoltre, il testo del provvedimento licenziato da ultimo alla Camera è privo di una norma, in precedenza con la quale si prevedeva che l'Agenzia per la sicurezza nucleare debba operare con indipendenza di giudizio, di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, con l'apporto di personale altamente qualificato. Perché è stata tolta questa previsione? A maggior ragione si rafforzano le nostre preoccupazioni circa l'inefficacia delle misure previste per garantire la sicurezza degli impianti nucleari. Il commissariamento della Sogin destava già perplessità in occasione del primo esame del provvedimento, perché riguarda una società che svolge il compito di provvedere al *decommissioning* degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi; il tutto in vista del conferimento delle medesime funzioni ad altre società di carattere privato e a partecipazione statale. Se da un punto di vista pratico temiamo che il prolungamento dei tempi del *decommissioning* possa far crescere gli oneri di smaltimento da trasferire a carico dei consumatori,

nel frattempo la Sogin rimarrebbe senza un organo che la governa. Il Gruppo del PD ha comunque contribuito alla stesura di questo testo per alcune parti. In particolare, si sono introdotte norme di fondamentale importanza per le imprese italiane, che lamentano l'onerosità dell'*iter* burocratico per ottenere autorizzazioni e concessioni. Infatti, è stata introdotta la previsione di una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, oltre alla previsione dell'autocertificazione come modalità attraverso cui alleggerire i procedimenti per l'ottenimento di titoli autorizzatori e concessori da parte della pubblica amministrazione. Quante volte, infatti, la pubblica amministrazione chiede alle imprese e ai cittadini certificazioni che magari riguardano atti o documenti già in suo possesso o comunque li costringe ad allungare i tempi del procedimento, che potrebbero essere ridotti se si introducesse con forza e convinzione il principio di autocertificazione? Sempre grazie al nostro contributo sono state introdotte misure importanti nel senso della trasparenza nella determinazione del prezzo di beni e servizi per i consumatori, come l'introduzione nel codice del consumo di una norma che stabilisce che è ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzino il prezzo del biglietto separatamente dagli oneri accessori o come la previsione di nuove forme di conoscibilità del prezzo dei carburanti, come quella della pubblicazione dei prezzi sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico. Abbiamo infine molto insistito sulla valorizzazione delle reti di impresa quale modello organizzativo che integra quello di distretto e lo può anche sostituire. infatti fa sì che ogni impresa possa mantenere la propria indipendenza ed individualità, che ne costituisce la forza, ma allo stesso tempo possa lavorare e collaborare insieme alle altre creando forme di organizzazione flessibile. Questo discorso vale ancora di più in questo particolare momento di crisi dei distretti industriali. Voglio dunque concludere il mio intervento auspicando che possa essere in qualche modo raggiunto l'obiettivo di dare maggiore omogeneità alle norme statali e regionali - per quello che riguarda le reti di impresa di carattere amministrativo, fiscale e finanziario, ed anche a quelle che riguardano la formazione e l'efficienza energetica, senza che vi siano contrasti e contrapposizioni o duplicazioni tra i diversi livelli.

Signor Presidente, come ha detto la senatrice Fioroni, questo disegno di legge da una parte mette al centro della politica energetica del nostro Paese l'inseguimento dell'opzione nucleare che, per come viene rappresentata, nasce tecnologicamente datata e si presenta con tali problematicità, in termini di costi economici, prima ancora che di accettazione sociale e di impatto ambientale, da configurarla come molto difficilmente realizzabile. Dall'altra, viene ulteriormente indebolito

che per le utenze di alta tensione. Ciò significa, molto concretamente, un grande aggravio di costi per alcune categorie di aziende, che oggi fanno cogenerazione. Cito, ad esempio, il caso delle cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione, che è ampiamente diffusa.

energetici sopportati dalle imprese e grandi vantaggi per l'intero Paese, visto che contribuisce ad alleggerire il peso della nostra bolletta energetica nazionale. In questo modo, invece, ci sono molte imprese italiane, soprattutto del settore manifatturiero, che vedrebbero caricata la loro produzione di energia in regime di cogenerazione di un aggravio che, soprattutto vista la crisi attuale, che durerà anche per i prossimi mesi, rischia di diventare per loro insopportabile. Nel momento in cui si sta aprendo all'Aquila il G8, nel quale uno dei temi all'ordine del giorno è quello di concertare tra i Paesi più ricchi e industrializzati del mondo scelte capaci di spingere all'innovazione energetica, in particolare in questo punto e non solo il disegno di legge che stiamo discutendo va nella direzione esattamente opposta. Mi auguro, se non altro,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, un giorno non si potrà certamente dire che questo provvedimento importante e vitale per l'economia e l'avvenire del nostro Paese non fosse stato sufficientemente delibato e discusso

Il provvedimento, pur passando ripetutamente al vaglio dell'esame parlamentare, non ha subito grandi modificazioni dall'epoca in cui lo abbiamo considerato e approvato. Ciò significa che, nonostante ogni migliore attenzione, poco c'era da rettificare, così come si è fatto. In questo provvedimento spicca il nuovo istituto delle reti di imprese, reti di imprese, che si rivelerà virtuoso e vitale per un'economia dove il 95 per cento è costituito da piccole e piccolissime imprese che, nonostante ogni migliore sforzo ed azione dei Governi del passato, non hanno conseguito il risultato pregevole della migliore commercializzazione dei loro prodotti proprio per effetto della polverizzazione del sistemo produttivo. Adesso, signor Ministro, noi guardiamo con molta attenzione e affidiamo a lei la disciplina e l'attuazione dell'istituto delle reti di imprese che certamente, se realizzato se realizzato appieno, dovrebbe consentire l'internazionalizzazione delle nostre microeconomie e, quindi, l'esaltazione del lavoro e della produzione dei cittadini italiani. Un'attenzione particolare avete pure riservato, onorevole Ministro, ai consorzi agrari. Questo è un grande istituto che per un lungo periodo è stato dimenticato nonostante nei decenni passati ci fosse stato invidiato da tutte le economie in via di sviluppo e fosse stato ritenuto il più grande istituto di ingegneria societaria mai pensato. L'averlo riconsiderato e rispolverato certamente ha dato soddisfazione a noi, che alla gente dei campi guardiamo sempre con grande rispetto e grande affetto. affetto. La SIMEST, se integrata dall'economia delle Regioni con i fondi rotativi previsti, potrà certamente esplicarsi e applicarsi su più vasta scala e all'estero dove ormai le nostre economie vanno a delocalizzare non anche per fuggire la Patria quanto per conseguire colà quelle economie che ormai - come mostra la teoria dei costi comparati e, in particolare, la comparazione del costo del lavoro di questo Paese con quello di altri in via di sviluppo - non ci consentono di poter avere i risultati che abbiamo avuto in passato.

La tutela della qualità delle produzioni, la tracciabilità, l'origine della stessa, l'attenzione che con la riconsiderazione dell'articolo lei ha voluto riservare alla pesca, completa questi due grandi ambiti a noi tanto cari dell'agricoltura e della pesca. L'AGEA,

il provvedimento sarà nelle sue mani tra poche ore e siamo fiduciosi che la sua competenza e la sua esperienza, onorevole Scajola, ci metteranno nelle condizioni di raccogliere nel breve periodo tutti i frutti che un disegno di legge così completo potrà dare al popolo italiano e alla sua economia.

validità o no dell'affrontare le tematiche dell'energia nucleare, che possono ben essere affrontate con una cultura peraltro assolutamente diversa, più moderna, aggiornata, quanto piuttosto sul tema della scelta dei territori su cui fare insistere le eventuali centrali nucleari,

dire l'avere affrontato il tema del federalismo per quanto soltanto sotto l'aspetto del federalismo fiscale e purtroppo non sotto quello più sostanziale del federalismo istituzionale. In questo senso credo che non si possa parlare di federalismo e quindi di esaltazione del ruolo delle autonomie locali e delle funzioni che le stesse devono esercitare per poi mortificarle di fatto nel momento in cui

in occasione della quale sono state date assicurazioni, con estrema certezza da parte di esponenti del Governo, secondo cui quella Regione sarebbe stata assolutamente immune dall'insediamento di centrali nucleari. Mi sarei aspettata a questo punto che un minimo di certezza potesse venire da un testo modificato dalla Camera dei deputati e che in realtà viene modificato in maniera improbabile negli effetti,

ad una sorta di vincolo di solidarietà nei confronti di altri territori nell'ambito di un discorso normale di unità nazionale. Ritengo però che quel *mix* energetico verso il quale pure l'Unione europea ci spinge ormai da anni e che è un dato ormai acquisito nella cultura comune debba, tuttavia, essere ponderato, voluto dai territori ed organizzato dalle istituzioni territoriali. territoriali. Le ripeto ancora una volta che, sia per espressione del Consiglio regionale sia per assicurazioni reiterate venute nella recente campagna elettorale dai vari rappresentanti del Governo - e lei sa che in Puglia abbiamo autorevoli

del territorio. Comprendo bene che le sto parlando semplicemente di una Regione, ma credo che se siamo eletti (o, meglio, nominati) da un territorio, quanto meno dobbiamo rispettare le esigenze dello stesso. Per questo motivo, Presidente, in assenza di un ordine del giorno che possa tranquillizzare realmente, ma soprattutto in carenza

Commento innanzitutto i pochi cambiamenti rispetto al testo approvato dal Senato subiti da questi tre articoli nel corso dell'esame alla Camera. Per quanto riguarda l'articolo 25, l'unico cambiamento è relativo alla lettera *n)* del comma 2. Nella versione approvata alla Camera viene semplicemente prevista la costituzione da parte dei produttori di energia nucleare di un fondo per il finanziamento del *decommissioning* a fine vita delle centrali. La definizione di *decommissioning*, non comparendo nelle definizioni delle leggi nazionali in materia, necessiterà di un chiarimento nell'ambito dei decreti delegati. Ragionando a buon senso, il fondo per il *decommissioning* dovrebbe coprire sia quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive sue modifiche, in riferimento alla parola disattivazione, che viene lì definita come «l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica», sia quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 368 del 2003 che prevede che «la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi rispetto delle condizioni in sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo, sia effettuata presso il Deposito Nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato». Nella versione approvata dal Senato si prevedeva inoltre che la gestione del fondo fosse attribuita agli stessi produttori che l'avrebbero costituito con i loro contributi. Sulla delicata questione di chi amministrerà il fondo per il *decommissioning* il disegno di legge al nostro esame non dice nulla, lasciando aperta al Governo qualunque possibilità di scelta. Per quanto riguarda l'articolo 26, la modifica introdotta dalla Camera al comma 1 riguarda la definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettronucleare realizzabili nel territorio nazionale. Non riguarda perciò assolutamente nulla di quanto ipotizzato dalla senatrice Poli Bortone un attimo fa. La delibera del CIPE prevista dal comma 1 per tale definizione dovrà essere adottata, ed è questa la novità introdotta dalla Camera, previo parere della Conferenza unificata permanente Stato-Regioni, che deve esprimersi entro 60 giorni. È effettivamente singolare che la Conferenza Stato-Regioni si esprima su una scelta avente caratteristiche sostanzialmente tecniche. L'impianto nucleare potrà essere del tipo EPR francese o del tipo AP1000 statunitense o di altri tipi ancora; le differenze di impatto sul territorio esistenti tra questi vari tipi d'impianto sono modeste. Per quanto riguarda l'articolo 29, la principale modifica apportata dalla Camera concerne il comma 3. In questo comma, nella versione approvata dal Senato, veniva garantita all'Agenzia per la sicurezza nucleare indipendenza di giudizio e di valutazione, piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare ed il riconoscimento della sua necessità di operare con personale qualificato ed altamente specializzato. Sono caratteristiche essenziali per il buon funzionamento di un'Agenzia per la sicurezza nucleare in qualunque Paese, come è evidente, e come prescrivono i regolamenti internazionali, ad esempio quelli della IAEA. L'esplicitazione di tali caratteristiche operative dell'Agenzia è stata soppressa nel testo approvato dalla Camera. È un passo non positivo, che comunque confidiamo non avrà alcuna influenza sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia non potrà non operare a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, se non con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia tecnico-scientifica e avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. E va sottolineata con chiarezza la seguente ovvietà: il buon funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è indispensabile per il ritorno del nucleare in Italia. Su di essa non si possono fare risparmi eccessivi. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi.

che tuttavia, per ovvi motivi, non possono essere apportati in questa occasione, data l'urgenza dell'approvazione del testo del disegno di legge al nostro esame, così come pervenuto approvato dalla Camera dei deputati. Tali miglioramenti sono i seguenti. al comma 2 dell'articolo 25 mi sarebbe sembrata opportuna l'introduzione tra i principi e i criteri direttivi della previsione di procedure trasparenti per pervenire alla scelta dell'ubicazione del deposito nazionale centralizzato dei rifiuti radioattivi ed alla definizione della sua struttura gestionale, coinvolgendo naturalmente le amministrazioni locali ed individuando chiaramente il regime di responsabilità nel medio e lungo periodo, come raccomandato dalle organizzazioni internazionali. La realizzazione del deposito nazionale centralizzato dei rifiuti radioattivi ha ormai assunto carattere di necessità urgente. Solo così potrà essere assicurata la gestione in piena sicurezza dei rifiuti radioattivi generati nel primo periodo di utilizzazione dell'energia nucleare nel nostro Paese. al riguardo segnalato che in base all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito in materia di riprocessamento (in Gran Bretagna) di combustibile nucleare irraggiato in Italia, il rientro nel nostro Paese dei prodotti radioattivi del riprocessamento dovrà avvenire entro il 2017. Un ulteriore successivo rientro in Italia di materiale radioattivo derivante dal riprocessamento di combustibile irraggiato a suo tempo avverrà nel 2025, in base all'accordo firmato in data 24 novembre 2006 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, riguardante il riprocessamento in Francia di tale combustibile nucleare. I tempi tecnici per la realizzazione del deposito nazionale centralizzato definitivo di rifiuti radioattivi a lunga emivita appaiono quindi ormai piuttosto stretti. Per quanto riguarda il principio e criterio *c*), di cui al comma 2 dell'articolo 25, mi chiedo francamente come possa pretendersi che i benefici diretti ai residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito siano caricati sulle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti elettronucleari, facendo divieto a tali imprese di trasferire gli oneri così determinati a carico degli utenti finali. Se questi oneri non saranno pagati dagli utenti finali da chi mai saranno pagati? Certamente non dai cittadini tramite imposizione fiscale. Così come è scritto, l'importantissimo principio e criterio direttivo *c*), essenziale per il ritorno al nucleare, mi sembra impraticabile. Circa l'articolo 25, comma 2, lettera *m*), c'è da chiedersi che cosa significhi «individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare per l'Agenzia dell'autorizzazione unica». Tali rischi sono difficilmente prevedibili. Non si vede come una società di assicurazione possa valutare questi rischi e offrire ai produttori strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa. Si pensa allora ad un contributo dello Stato, parziale o totale, a copertura di questi rischi? In effetti, negli USA con l'*Energy Policy Act* del 2005 è stata prevista da parte dello Stato la copertura di eventuali perdite dovute a ritardi nella costruzione (non imputabili alle imprese) fino ad un ammontare massimo di 500 milioni di dollari per le prime due centrali nucleari e fino a 250 milioni dalla terza alla sesta centrale. Anche in Francia è lo Stato a coprire direttamente i rischi di danni conseguenti a ritardi non imputabili agli operatori, estendendo, attraverso la COFACE, la copertura dei rischi di questo tipo alla costruzione di centrali nucleari all'estero. Come si vede, le uniche esperienze finora esistenti di copertura assicurativa e finanziaria dei rischi a cui sono esposti i produttori di energia elettronucleare prevedono che sia lo Stato ad effettuare la suddetta copertura. Se tale forma di assicurazione pubblica dovesse essere adottata anche in Italia, si porrebbe ovviamente un problema di copertura dei relativi oneri nel bilancio dello Stato; tuttavia, tale copertura non è stata prevista nel disegno di legge Sempre al comma 5 dell'articolo 29, alla lettera *i*), riterrei più opportuna la parola «approva» al posto della parola «definisce». Infatti i soli che dispongono di tutte le informazioni necessarie per definire nel dettaglio le procedure per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento degli impianti a fine vita sono i titolari autorizzati all'esercizio o allo smantellamento. L'Agenzia per la sicurezza nucleare è in grado di definire non le procedure, ma le linee guida per le stesse ed in ogni caso ad essa compete la loro approvazione. In conclusione, conclusione, con l'imminente approvazione del disegno di legge al nostro esame si compie il primo fondamentale passo per la reintroduzione nel nostro Paese dell'energia nucleare, un obiettivo assai complesso, di grande rilevanza simbolica ed economica, che il Governo Berlusconi ha saputo coraggiosamente assumere all'indomani della vittoria nelle elezioni politiche dell'aprile 2008. Il prossimo passo competerà al Governo con la creazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'elaborazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 25. Auguri cordiali di buon lavoro!

perlomeno si discuta di nucleare, visto che dopo la nostra votazione sarà tutto solo ed esclusivamente nelle mani del Governo. Non c'è nessun pregiudizio, né alcun preconcetto che sta alla base della nostra contrarietà al provvedimento in esame, in particolare per la parte riguardante il nucleare e, appunto, la delega al Governo, su cui vorrei però soffermarmi. Alle richieste di confronto che da oltre un anno stiamo avanzando (e parlo soprattutto come delegazione radicale nel Gruppo del PD), alle perplessità che la scelta del nucleare sia quella più conveniente, nessuna risposta; solo annunci propagandistici e misure illiberali che impongono scelte, impedendo un confronto su costi e benefici.

La tipologia degli impianti sarà decisa dal CIPE; per costruirli e farli funzionare basterà un'unica autorizzazione che verrà rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, d'accordo con i colleghi dei Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture: una partita di giro all'interno di Palazzo Chigi. Si istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, composta da un presidente e da quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, anche in questo caso senza neppure dare la parvenza che sia un'Agenzia indipendente. In pratica, il Governo chiede ed esige un mandato in carta bianca, per fare come meglio crede, senza bisogno di consultare il Parlamento, né tanto meno gli enti locali: alla faccia del federalismo! Non è un caso che il nucleare è fermo da tempo là dove le preoccupazioni e il controllo dell'opinione pubblica hanno più peso e dove l'energia è un affare di mercato; invece continua ad andare avanti in Cina, in India, in Russia, dove il controllo democratico o non c'è, oppure è molto più fragile e dove le centrali vengono pagate con i soldi dello Stato. Nel complesso il nucleare è in declino l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) calcola che nel 2030 la quota di elettricità prodotta nelle centrali atomiche si ridurrà dall'attuale 16 al 9-12 Si dice però che la scelta del nucleare serva a diminuire la nostra dipendenza da fonti energetiche (petrolio) dall'estero: è un falso, e vediamo perché. la tecnologia nucleare è di importazione francese e la Francia, con il suo 78 per cento di produzione elettrica nucleare, consuma più petrolio della Germania: se è vero che la Francia ci vende energia elettrica nelle ore morte, (è sovracapacitata), nelle ore di punta la compra dalla stessa Germania. Il combustibile l'uranio, è estero: il 58 per cento delle riserve sono in Canada, Australia e Kazakistan. Il premio Nobel Carlo Rubbia già ci mette in guardia sulla poca disponibilità dell'uranio a livello mondiale e di conseguenza il prezzo dello stesso è soggetto a speculazioni, come come e peggio del petrolio. Se la dinamica sarà la stessa che l'uranio ha seguito dal 2000 ad oggi, aumentando di venti volte da 7 a 130 dollari per libbra (ha spiegato così il fisico premio Nobel), il prezzo potrebbe arrivare anche a 500 dollari e il costo dell'elettricità nucleare schizzerebbe da 40 a 65 euro per megawatt, un livello insostenibile. Si aggiunga il problema della disponibilità: le riserve conosciute valgono per non più di una trentina d'anni; per due terzi il mercato dipende dalle forniture militari il più grande impianto di estrazione, quello di Cigar Lake in Canada, tarda ad entrare in esercizio. Ancora, tra i vantaggi di questa scelta ci si dice che «il nucleare dovrà produrre un quarto dell'energia elettrica del Paese (25 per si finge di dimenticare che la produzione elettrica italiana rappresenta il 18 per cento del nostro fabbisogno energetico complessivo, l'82 per cento del quale (carburanti e così via) va essenzialmente ai trasporti. l'obiettivo del 25 per cento del ministro Scajola, rispetto al 18 di produzione elettrica, significa che il nucleare sarà il 4,5 per cento del fabbisogno di energia elettrica. cento, l'alternativa c'è già, ed è quella di puntare sull'efficienza energetica, la più grande fonte di energia a detta di tutti gli esperti. Ciò significa evitare gli sprechi. La via è quella di un *mix* di energie rinnovabili: efficienza energetica, solare, eolico e quant'altro la tecnologia odierna possa offrire. E poi la ricerca. Un recente studio dell'istituto McKinsey, uno dei più accreditati a livello mondiale, spiega come con l'efficienza energetica nella costruzione di edifici si possa coprire il 4 per cento del nostro consumo nazionale: la stessa cifra delle centrali nucleari. sarebbe la strada da percorrere, sembra abbastanza ovvio; lo si può fare da subito e spendendo molto meno. Infine, non possiamo non porci il problema, tutt'altro che marginale, della sicurezza e delle scorie, tra l'altro in un Paese in cui non si riesce neppure a smaltire la spazzatura. Dopo il *referendum* del 1987, non siamo ancora riusciti, nel 2009, a liberarci delle vecchie scorie stoccate in luoghi non adatti, come a Saluggia,

ci lanciamo in questo passo - con un ritorno al passato, un tuffo all'indietro - del nucleare. Senza un piano energetico nazionale non si vede davvero che tipo di politica si possa e si intenda programmare; senza tale piano, le date e le cifre di cui parliamo le cifre di cui parliamo restano solo dei numeri che non hanno alcun senso. Signor Presidente, in un intervento precedente si è detto, cogliendo una verità, che oggi il mondo ci guarda. è vero, ma potremmo anche aggiungere che oggi il mondo, a guardarci, sorriderebbe nel verificare ciò che stiamo approvando in materia di energia.

assolutamente non comprensibili dal punto di vista di una visione politica ottimale. Siamo il Paese

Mentre nel resto del mondo i concessionari dei pozzi di estrazione pagano

che non vanno a beneficio dello Stato a discapito del territorio su cui insistono i pozzi estrattivi; è denaro, invece, dato in beneficio ai concessionari, cioè a coloro che hanno ottenuto la concessione di perforare il nostro territorio estraendo energia e idrocarburi liquidi o gassosi. E penso alla mia Regione:

L'aumento che il Governo ha deciso con questo provvedimento porta dal 7 al 10 per cento l'aliquota che devono pagare i concessionari, ma non per i pozzi a mare, ossia quelli che rientrano nel mare della mia Provincia. Sono decine e decine di milioni di euro, che, in base alla legge, vanno in parte allo Stato e in parte al territorio: è un furto, che si consente nonostante il nostro sforzo di chiedere una modifica radicale nella direzione di un adeguamento del pagamento delle cosiddette *royalties*,

ed ora lievemente aumentate al 10 per cento. Non conosciamo la ragione per cui il Governo non voglia ridare i benefici economici ai territori che offrono questo prodotto, il cui lucro è è garantito solo ai concessionari. Questo poteva spiegarsi forse quando i concessionari erano pubblici, ma ora sono privati: perché non devono pagarci il prodotto e dobbiamo regalarglielo? Perché il resto del mondo garantisce i territori e noi no? Il secondo punto che qualifica questo provvedimento è l'opzione netta

fatta dal Governo con la previsione della realizzazione delle centrali nucleari di terza generazione,

saranno realizzabili le centrali nucleari di quarta generazione. Questo significa che di qui a dieci o dodici anni andremo a realizzare centrali nucleari con un sistema rischioso e sorpassato,

senza considerare che rimane ancora insoluto, a livello mondiale, il problema del trattamento delle scorie.

25.000 metri cubi di rifiuti di combustibile irraggiato, cui si sommano 1.500 metri cubi prodotti annualmente dai settori della ricerca, e 80.000-90.000 metri cubi derivanti dallo smantellamento delle quattro centrali. Ancora non abbiamo risolto questo problema, ben sapendo che tutti gli studi certificano che il trattamento delle scorie attualmente in atto (ossia la cosiddetta vetrificazione) è garantito per non più di 100 anni. Ciò significa che il trattamento di vetrificazione non riuscirà a contenere le scorie. Il nostro pianeta ha tante bombe atomiche disseminate. Non riusciamo ad eliminare le scorie e ci avventuriamo verso la strada del nucleare, che è abbandonata dal resto del mondo. Non riusciamo a cogliere le ragioni politiche, se non attraverso una interpretazione lobbistica di queste scelte. che mentre nel resto del mondo si va avanti verso le energie alternative, noi abbandoniamo la strada delle energie alternative, quelle che nel resto del mondo si stanno sfruttando alle conoscenze e alle industrie italiane: e in Italia no! Dovete spiegarci il perché di tutto ciò. Perché le nostre industrie possono realizzare gli impianti in Spagna, in Libia, nel Nevada e non in Italia?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è stato predisposto per affrontare alcune problematiche di natura strutturale che investono importanti settori strategici dell'economia del nostro Paese e che, di fatto, impediscono al nostro sistema produttivo di emergere da una situazione di generalizzato stallo economico. Gli argomenti affrontati sono sostanzialmente tre: sviluppo delle piccole imprese e del commercio internazionale, tutela della proprietà industriale e lotta lotta alla contraffazione e adozione di nuove strategie energetiche nazionali, con il riassetto di importanti enti che operano nel settore. Il tema dell'energia, come tutti sappiamo,

politiche ecologiche, investimenti di valorizzazione delle fonti di produzione delle energie rinnovabili, sia industriali che agricole. Con questo provvedimento viene incentivata per il mondo agricolo la realizzazione di impianti a biomassa non molto grandi, di ridotte dimensioni, quindi facilmente realizzabili in molte aziende agricole, con potenze inferiori a un megawatt. Ciò offrirà certamente nuove possibilità di far impresa e sarà fonte di reddito per gli agricoltori che potranno integrare e diversificare le attività dell'azienda nell'ottica di un'agricoltura sostenibile, sia dal punto di vista energetico che ambientale. In questo provvedimento viene affrontato anche il tema della trasparenza dei prodotti alimentari. Troviamo espressamente, all'articolo 17, un'anticipazione di quello che presto sarà un provvedimento che il Governo, tramite il Ministro dell'agricoltura, attuerà, presentando in maniera più organica e complessa l'etichettatura, cioè la tracciabilità dei prodotti agricoli, a tutela della salute dei consumatori. In questo provvedimento si regolamenta l'identificazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, andando finalmente nella direzione della tutela e dell'informazione del consumatore, attraverso l'obbligatorietà dell'esposizione di tantissime informazioni sull'etichetta dei prodotti ittici.

di qualità e di genuinità del prodotto ittico venduto all'interno del nostro Paese. Energia pulita, rinnovabile, a buon mercato, ecologicamente sostenibile: è con questa filosofia che all'articolo 27 di questo provvedimento - grazie ad un emendamento proposto dalla Lega Nord - abbiamo dato la possibilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti

gli impianti di potenza fino a 20 kilowatt ed estendendo chiaramente i benefìci per lo scambio sul posto, che oggi è in vigore per impianti fino a 20 kilowatt, a tutto il territorio comunale per gli impianti fino a 200 kilowatt. Diamo quindi la possibilità ai Comuni medio-piccoli, che hanno una popolazione di circa 4.000-5.000 abitanti, di produrre l'energia elettrica di cui hanno bisogno per le esigenze delle proprie utenze. Non serve molto spazio per poterlo fare: bastano circa

nostro esame, nel suo insieme, ci permetterà certamente di dare nuovo slancio all'economia e di recuperare quel *gap* energetico che, negli ultimi anni, aveva visto il nostro Paese particolarmente arretrato nei confronti dei Paesi più all'avanguardia. È per questo che il movimento della Lega Nord voterà con convinzione a favore di questo provvedimento.

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, torna nell'Aula del Senato, in quarta lettura, questo provvedimento a circa un anno dalla sua adozione in Consiglio dei ministri e dopo che ha conosciuto un progressivo stravolgimento ed ampliamento nel merito delle questioni trattate e nella dimensione del testo, passato da 17 articoli iniziali a ben 64. Torna in quest'Aula, dopo l'ulteriore esame da parte della Camera, un testo che avremmo voluto e sperato fosse migliore di quello licenziato dal Senato circa due mesi fa e che invece, proprio per via di alcune delle modifiche apportate, ci ritorna purtroppo, per alcuni aspetti, peggiorato. Siamo di fronte, infatti, ad un testo che lascia innanzitutto irrisolti alcuni gravi limiti che nel corso del lungo esame in Senato abbiamo evidenziato con forza e che hanno indotto il Gruppo del Partito Democratico a votare contro, sia alla Camera che al Senato, il provvedimento nel suo insieme: dal sostanziale svuotamento della norma sulla *class action*, tanto attesa dal mondo dei consumatori, che rende pressoché impraticabile l'azione risarcitoria collettiva, all'incomprensibile, per molti aspetti, maxiemendamento di un collega senatore della maggioranza con cui si è modificata la legislazione sul trasporto ferroviario nel nostro Paese, un maxiemendamento che, per ampiezza, specificità e contenuti si è configurato come una sorta di provvedimento nel provvedimento; e ancora, all'arretramento sul terreno delle liberalizzazioni e della tutela dei consumatori, che si è manifestato nel settore delle assicurazioni, l'introduzione dell'impossibilità, per gli assicurati attraverso polizze poliennali, del recesso anticipato: un regalo - chiamiamolo con il proprio nome - alla potente *lobby* delle assicurazioni nell'ambito di un articolo del disegno di legge in questione, che recita testualmente: «Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi»; ebbene, giudichi ognuno di voi, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Presidente, la coerenza tra la rubrica di questo articolo e il merito; il merito; per finire con il corposo capitolo del cosiddetto ritorno al nucleare che, da parte nostra, abbiamo affrontato in questi mesi, al contrario di vasti settori del Governo e della stessa maggioranza, senza alcun pregiudizio di natura ideologica. che il nucleare è questione troppo seria per essere affrontata in termini ideologici. Abbiamo avuto modo di denunciare, negli scorsi mesi, la forzatura con cui, nel pieno dell'*iter* parlamentare di un provvedimento che concerne una materia così delicata, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa - e il ministro Scajola lo ricorda bene - tra il Governo italiano e quello francese che, in qualche modo, prefigura quelli che saranno, una volta che tale provvedimento diventerà legge, i requisiti e le tipologie degli impianti che verranno utilizzati nel nostro Paese, attraverso un rapporto privilegiato con l'industria francese. Sostanzialmente, stiamo cedendo una parte del mercato energetico italiano ad una tecnologia ormai obsoleta, rinunciando alla sollecitazione di un'adeguata competizione internazionale, che non si potrà realizzare a causa dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e il Governo francese, tra l'ENEL e l'EDF. Di questo stiamo parlando. Così come non possiamo non tornare a denunciare le forzature delle procedure, specie nel rapporto democratico con le comunità locali e con le istituzioni locali, chiamate alla espressione di un mero parere consultivo e non, invece, vincolante, come abbiamo proposto con i nostri emendamenti, bocciati sia alla Camera che al Senato, per la definizione dei decreti delegati che andranno a regolamentare la scelta dei siti, delle tipologie di impianti, dei processi di smaltimento delle scorie e così via. In realtà, non solo non si è messo mano a tali aspetti negativi, che abbiamo provato ad alleviare con i nostri emendamenti, prima in Senato e poi alla Camera, ma il testo che torna qui oggi, seppur modificato in punti assolutamente parziali, ha il segno di un ulteriore peggioramento. Penso all'articolo 1, che definisce le disposizioni per la operatività delle reti di impresa, terreno su cui si è consumato un altro capitolo di una guerra - mi perdonerà il ministro Scajola - non tanto sotterranea, di competenze e primazia tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico, che vede, purtroppo, soccombere quest'ultimo a seguito delle modifiche introdotte, che capovolgono la competenza nell'emanazione di alcuni decreti attuativi a vantaggio, appunto, del Dicastero Penso all'articolo 25, che definisce l'ambito della delega al Governo in materia di energia nucleare e i principi che devono ispirarne il concreto esercizio: qui si consuma, infatti, un altro grave strappo, cancellando, peraltro, una norma introdotta proprio qui, in Senato. Mi riferisco alla previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning*, per il quale viene soppresso il vincolo a che tale fondo sia esplicitamente costituito con una contribuzione a carico dei produttori medesimi, come espressamente richiamato nel testo licenziato dal Senato unitamente alla previsione, anche questa soppressa, che tali risorse potevano essere attribuite agli enti locali che ospitano gli impianti. Mi sembra un arretramento del tutto evidente. Per concludere, richiamo altre due modifiche: all'articolo 27 cui, quasi in una sorta di accanimento, si prevede che la decadenza degli organi amministrativi della Sogin avvenga non più alla data di nomina dei commissari straordinari, ma alla data di entrata in vigore della presente legge, con il rischio, evidentemente, di un periodo di assenza di guida e di confusione gestionale di una così importante e delicata struttura.

il seguente periodo: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato». una norma che garantiva la terzietà, l'autonomia e la qualità di un organismo chiamato a compiti straordinariamente delicati, che ora con un tratto di gomma vengono cancellate. Il nostro Gruppo ha inteso presentare pochi ma significativi emendamenti e alcuni ordini del giorno sulla parte modificata del testo, che vanno nella direzione di ripristinare i testi precedenti, peggiorati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, nonché di migliorare quelle garanzie, che sono state affievolite, di di terzietà e di affidabilità delle strutture la cui funzione è assolutamente delicata. Mi auguro che il Governo e la maggioranza colgano il senso di collaborazione che viene dalle proposte del Partito Democratico e possano accoglierle come meritano, nell'interesse del Paese.

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1195-B rappresenta una risposta concreta del Ministro, del Governo e anche del Parlamento a due esigenze fondamentali dello sviluppo del Paese: lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e l'energia.

in particolare quelle piccole e medie. Sono diversi i fattori significativi che troviamo come elementi in favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione delle imprese e in particolare, come dicevo, delle piccole e medie imprese: vanno tutti nel senso di offrire strumenti di aggregazione, di semplificazione amministrativa, di miglioramento della conoscenza e di sviluppo della concorrenza internazionale. Il primo elemento è rappresentato senz'altro dallo strumento della rete di imprese, ovvero dall'aggregazione tra piccole e medie imprese, anche distribuite in diverse zone del Paese, sulla base di progetti comuni. In questo modo le piccole e medie imprese, senza perdere la propria identità e la propria efficienza, possono ampliare il proprio mercato, avendo a disposizione strumenti per migliorare l'economia di scala ed il livello dell'innovazione e della conoscenza, ottimizzando altresì, eventualmente, anche i processi di produzione. L'evoluzione informatica consente sempre di più di considerare l'aggregazione di imprese non solo su scala di particolari ambiti territoriali, come avvenne per i distretti produttivi, dove molto spesso l'aggregazione non è stata tanto per prodotto/processo produttivo, cioè non tanto per "progetto", ma per la messa in comune di servizi e di infrastrutture. La rete di imprese, così come viene chiaramente definita, si basa quindi non sul concetto di "aggregazione territoriale", ma particolarmente su "aggregazione su progetto", che rappresenta una grande evoluzione, ed ha quindi maggiore potenzialità di incrementare la ricerca e l'innovazione, aprirsi verso i mercati internazionali, sfuggire ad un'influenza politica e sindacale a volte troppo presente sia nei distretti che nelle grandi imprese, migliorare il proprio sistema di impresa traendo vantaggio dal confronto con le altre facenti parte della rete ed incrementare la propria partecipazione ai progetti europei, ampliando eventualmente la rete anche ad imprese estere. Come si vede, si tratta quindi di elementi estremamente significativi. L'emendamento da me presentato e già approvato in Senato, condiviso anche da gran parte dell'opposizione, introduce nell'articolo 1 l'estensione di vantaggi e agevolazioni, riservati fino ad oggi solo ai distretti industriali, industriali, anche alle reti di imprese, consentendo all'Italia un salto in avanti verso la competitività. Nel testo che stiamo discutendo si definisce, quindi, per la prima volta in maniera dettagliata il contratto di rete, con il quale due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Non elenco tutti gli elementi che sono parte integrante del contratto che viene redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Desidero menzionare soltanto uno di questi punti, che è estremamente importante: questo contratto richiede l'individuazione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune. inoltre, un organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, portando su una centralità di tipo manageriale e gestionale le imprese che afferiscono alla rete di imprese.

Si ricorda che il comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha recato numerose disposizioni per i distretti produttivi che, come dicevo prima, vengono ampliate al concetto di reti di imprese.

amministrative e di ricerca e innovazione, previste precedentemente solo per le imprese all'interno dei distretti, noi mettiamo in condizione le piccole e medie imprese di aggregarsi su scala nazionale ed internazionale per affrontare meglio il mercato.

di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale. Dato il tempo ristretto non menziono altri punti, desidero mettere in risalto che la lungimiranza di questa legge comporta al proprio interno altri elementi significativi che favoriscono la piccola e media impresa - che, come si sa, è la struttura portante del nostro sistema industriale nazionale

Dall'altra parte, sono presenti tutti gli elementi tesi a promuovere i rapporti con l'estero grazie all'attivazione di misure per lo sviluppo del *made in Italy*, per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio. Ora, nella semplificazione normativa, si deve tener conto di alcuni temi importanti tra cui, ad esempio, quello della semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni, oltre alla differenziazione e alla regolamentazione delle misure di incentivazione, ove necessario, in funzione della dimensione dell'intervento agevolato ovvero dei settori economici di riferimento. un lato, prevale dunque un concetto di sviluppo di rete di impresa, che crea una grande potenzialità per le piccole e medie imprese in termini di aggregazione per progetto e per finalità di produzione e di innovazione; dall'altro, si riporta nell'ambito delle piccole e medie imprese, e quindi della rete di impresa, una serie di opportunità, derivanti dalla semplificazione normativa, di incentivazione per l'innovazione e la ricerca, per l'internazionalizzazione, e menzionerei anche la lotta alla contraffazione e il diritto industriale.

Queste, con l'intelligenza e l'impegno che le caratterizza, sapranno cogliere pienamente le opportunità offerte per crescere e svilupparsi, opponendo efficienza e conoscenza

che, con lettera in data 8 luglio 2009, il senatore Giovanni Collino ha dichiarato, a seguito della propria elezione a parlamentare europeo, di voler rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica, con decorrenza dalla prima seduta del Parlamento europeo, che avrà luogo il 14 luglio 2009. Trattandosi di dimissioni originate da motivi di incompatibilità e conseguenti ad un'opzione, quest'Assemblea non può che prenderne atto. Pertanto, le dimissioni dispiegheranno effetto a partire dal 14 luglio 2009. Collega Collino, questa Presidenza intende darle atto del lavoro svolto e farle anche i migliori auguri per il lavoro che

Colgo l'occasione per ringraziare della collaborazione i membri del Governo e tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. La mia elezione al Parlamento europeo non era prevista.

Cercherò di fare del mio meglio, con serietà ed abnegazione, per rappresentare l'Italia nel Parlamento europeo. *(Generali

Signor Presidente, onorevoli Senatori, ho seguito con attenzione l'andamento della discussione generale e le posizioni espresse dagli esponenti della maggioranza e delle opposizioni. Al di là delle diverse valutazioni, credo che sia chiara a tutti la rilevanza strategica del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare: possiamo affermare che con questo provvedimento passiamo dalle misure di emergenza per contrastare la crisi a riforme strutturali per aiutare il Paese e il sistema produttivo ad uscire dalle attuali difficoltà, avviando processi di competitività,

e per permettere una celere approvazione di questa importante legge, onorevoli colleghi, consegnerò il testo del mio intervento alla Presidenza perché possa essere

lettura dei pareri della 5a e della 1a Commissione apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 25.3 e 29.5, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la disciplina organica dei canoni minerari e delle aliquote di prodotto che

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

la Provincia dell'Aquila e per i Comuni del cratere, è occasionata dall'esistenza in questo provvedimento di una norma che riattribuisce risorse finanziarie certe alle zone franche urbane così come erano state istituite e regolamentate nella finanziaria per

la possibilità di istituire in quei territori disastrati zone franche urbane - fu ritenuta necessaria sia da parte nostra che della maggioranza,

con una somma di 45 milioni di euro per il 2009, lasciando impregiudicata la possibilità, (direi la necessità) di finanziare per gli anni successivi le importo di eguale entità. Tant'è che noi presentammo sia in Commissione che in Aula emendamenti volti ad estendere la copertura anche al triennio successivo. Se nonché il Governo in Aula, a conclusione dell'esame del provvedimento, presentò un suo emendamento volto a modificare la norma che era stata approvata dalla Commissione, stabilendo che

cioè poco più di 10 milioni di euro all'anno, una cifra che definire insufficiente è eufemistico: si tratta di una cifra larghissimamente insufficiente a far fronte a qualunque esigenza di quei territori.

la zona franca urbana a tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila, come avevamo già proposto in Commissione, oltre che ai pochi altri Comuni del cratere situati

di forte incentivazione e di forte attrazione degli investimenti, seppure riferiti a piccole attività economiche, ma rappresentano oggettivamente un elemento distorsivo della concorrenza. È evidente che, se si incentiva con una

si estenda all'intero territorio interessato questo tipo di misura incentivante. del 2009 non ci sono, come è noto, altre risposte significative per far riprendere le attività economiche in quei territori. Ne abbiamo già discusso e non è questa la sede per riproporre quegli argomenti, ma ciò che noi prevedevamo, e cioè che la struttura di quel decreto e in particolare il fatto che non fossero in esso individuate misure precise a sostegno dell'economia costituisse un gravissimo limite del provvedimento stesso, si sta puntualmente verificando.

all'esame della Camera, il Governo ha addirittura stabilito che, a partire da gennaio del prossimo anno, dovranno essere restituite le imposte sospese a seguito dell'emanazione delle ordinanze,

all'Aquila costituisce una straordinaria vetrina, un'occasione, ma come qualunque occasione la si può cogliere oppure no. E io temo - tutti temiamo - che, spenti i riflettori del G8, si spegneranno anche i riflettori dell'attenzione sui sui gravissimi problemi che le aree terremotate stanno vivendo in queste settimane. Le proposte che formuliamo sono assolutamente ragionevoli. La copertura finanziaria è garantita, poiché si attinge al Fondo strategico per il Paese che in parte consistente è già destinato a finanziare gli interventi per la ricostruzione. Sarebbe una buona notizia se l'Aula del Senato accogliesse oggi queste proposte emendative necessarie ed assolutamente ragionevoli. Sollecitiamo un'apertura in questo senso da parte del Governo e speriamo vi sia sensibilità da parte dei colleghi

a tale problematica. Il nostro timore, ripeto, è che dopo il G8 tutto passi sotto silenzio e che le sofferenze e i problemi non risolti di quei territori siano destinati ad accrescersi. Le preoccupazioni

La ricostruzione ancora non parte, l'economia non sta ripartendo. Occorrono misure urgenti, e questa è una misura assolutamente necessaria per riavviare per riavviare l'economia di quei territori. Ecco perché confidiamo nell'attenzione e nel voto favorevole dei colleghi della maggioranza.

In particolar modo lo chiede ai senatori abruzzesi di questa Assemblea, che sanno benissimo in quali condizioni si trovi l'economia reale di quella terra e conoscono benissimo i problemi derivanti dal danno diretto ed indiretto provocato dal sisma del 6 aprile Lo sanno perché sono a conoscenza di tali problemi, anche se il loro spirito di giusta devozione alla maggioranza li porta a non rompere con la loro maggioranza e con il Governo. Vi chiediamo, senatori abruzzesi, di collaborare affinché le imprese, l'economia, il lavoro, l'occupazione che non sono stati tutelati dal decreto‑legge n. 39, ora diventato legge dello Stato, possano avere con gli emendamenti in esame la giusta attenzione che oggi, come voi sapete, non hanno. Vi chiediamo, colleghi, di ragionare su questo punto: non ci sono forzature, non ci sono spese inutili, non stiamo allargando l'intervento dove il danno non c'è stato. Stiamo intervenendo su Comuni, su realtà imprenditoriali, su luoghi di lavoro che hanno subito danni

oggi in quest'Aula questi due emendamenti o anche uno di essi. Il presidente Berlusconi potrebbe dire, di fronte ai Grandi della Terra, che grazie al voto unanime di questo Parlamento e della sua maggioranza ha portato per tutta quella terra un risultato incredibile, proprio in questa giornata.

anche quello che di vero c'è in questa situazione e in questa terra. Un'attenzione che non abbiamo ricevuto dal Governo e un no pregiudiziale, inizialmente

per porre rimedio ad un problema non risolto nel vostro decreto-legge, ora diventato legge dello Stato. Vi chiediamo di appoggiare questa proposta

Presidente, in questo secondo emendamento, a differenza del primo, si dà certezza

è precisato che per la costituzione delle zone franche urbane si possono spendere fino a 45 milioni di euro. C'è scritto che "si possono" spendere, il che vuol dire che è anche possibile non spendere e quindi non utilizzare quelle somme. Il secondo aspetto da rilevare è che, nello stesso emendamento presentato dal Governo,

la realizzazione di zone franche urbane nell'ambito del procedimento di approvazione europea. Il Partito Democratico chiede ai colleghi dell'Assemblea di appoggiare questo emendamento e, ancora una volta, chiedo ai senatori abruzzesi di sottoscriverlo e di votarlo tutti insieme, per il bene degli abruzzesi.

In particolare, è stata modificata la lettera *n)* sopprimendo le disposizioni introdotte dal Senato nelle quali si esplicitavano le finalità del fondo di *decommissioning*.

Signora Presidente, l'emendamento 25.2 ha l'obiettivo di reintrodurre la formulazione con cui questo testo era stato licenziato dal Senato con riguardo al fondo per il *decommissioning* degli impianti per l'energia nucleare. la formulazione è stata quasi del tutto cancellata; in questo modo, in particolare, non si prevede più che le risorse finanziare di cui al fondo per il *decommissioning* possano essere attribuire, oltre che alla Provincia e al Comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai Comuni confinanti. Visto che, come tutti sanno, generalmente gli impianti per la produzione di energia nucleare sorgono di Comuni di non grandi dimensioni e le problematiche collegate hanno un impatto anche sui Comuni confinanti, credo che la cancellazione di queste disposizioni rappresenti un fatto molto grave, destinato ad accrescere le preoccupazioni delle comunità

il Governo a predisporre, nell'ambito della "Strategia energetica nazionale" da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico così come previsto dall'articolo 7 della legge n. un piano dettagliato sugli interventi in materia di energia nucleare che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto. Il piano sarà illustrato al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione del DPCM che definisce la "Strategia energetica nazionale"».

mentre i primi punti manterrebbero la loro qualificazione di ordine del giorno, per l'ultimo punto accettiamo che venga accolto come raccomandazione.

si rimette al Governo

e in realtà sul complesso della proposta che formulano il Governo e la maggioranza in materia di

Una sola volta, nel 2007, abbiamo raggiunto il 60 per cento di produzione energetica. Per di più, la delega presuppone il fatto che si travalichi il rapporto tra Stato, enti locali e territori: l'individuazione di siti strategici nazionali, anche se con un passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, toglie infatti totalmente la possibilità di concertare i luoghi di insediamento delle centrali. Faccio notare che nel nostro Paese non c'è un solo luogo, se non le coste, dove esiste una quantità di acqua sufficiente a raffreddare le centrali nucleari. Non siamo in condizione di farlo nella Pianura padana e dovremo quindi scegliere le coste.

assunta dalle popolazioni (al contrario di quanto questo disegno di legge presuppone), come un fatto favorevole. Se escludiamo la Puglia, la Sardegna

Devo ancora dire che una delega che rimette totalmente nelle mani dell'ENEL e dell'accordo tra l'ENEL e la Francia l'adozione di centrali nucleari francesi di terza generazione,

seguendo le traiettorie del nucleare di quarta generazione e cercando di patrimonializzare quel poco o molto che è rimasto all'industria energetica nazionale riguardo alla capacità di progettare e proporre innovazione in materia.

questi articoli siano di puro orientamento propagandistico, che non avranno mai alcun senso attuativo. Con una spesa di questo genere si potrebbe finanziare per 100 volte la ricerca nucleare di quarta generazione. si punta su sistemi tecnologici che in moltissimi altri Paesi sono ormai considerati del tutto obsoleti: ricordo che negli Stati Uniti dal 1972 non si costruiscono centrali nucleari di questo tipo. condizionato dalla paura o ideologicamente contrario al nucleare, ma per dimostrare che vi è una totale inadeguatezza di progetto industriale sul nucleare italiano e una totale inadeguatezza di tipo economico di questo intervento. Spendere per centrali nucleari mentre abbiamo un *surplus* di produzione energetica vuol dire che l'investimento strutturale ricadrà come ammortamento sulla bolletta energetica nazionale dei contribuenti;

non aumenta la nostra indipendenza dal punto di vista dei combustibili, perché l'uranio è un combustibile limitato, per cui siamo totalmente dipendenti dall'estero, mentre il nucleare di quarta generazione ci consente di utilizzare le scorie, di impiegare più ricerca e più industria italiana e di avere minori problemi di approvvigionamento. Francamente, se molti dicono che non vi sono le ragioni di sicurezza, io sostengo, credo consapevolmente, che non vi sono né le ragioni scientifiche, né le ragioni industriali, né le ragioni economiche per essere favorevoli a una delega sul nucleare, in questo momento, nel nostro Paese.

Presidente, noi proponiamo di arricchire l'articolo 26 rendendo più significativa la partecipazione delle Regioni e degli enti locali. Il CIPE delibera circa la scelta delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, che devono poi essere realizzati sul territorio nazionale, comportando con questa decisione un coinvolgimento diretto nell'ambito delle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali. Alla Camera è stato accettato l'emendamento che prevede il parere della Conferenza unificata, ma quel parere, secondo la nostra valutazione, deve essere assegnato un tempo congruo perché la Conferenza unificata possa esprimersi in ordine alle tecnologie che si pensa di impiegare. Per questo motivo chiediamo

delle istituzioni locali, noi siamo convinti che il percorso che proponiamo possa risultare più in grado di determinare le condizioni attraverso le quali

questioni delle quali le Regioni e gli enti locali sono titolari. Per questo chiediamo di considerare con attenzione questi emendamenti sui quali ovviamente noi ci esprimeremo positivamente.

il coinvolgimento delle comunità locali e delle loro istituzioni, Comuni, Province e Regioni, in particolare attraverso lo strumento e la sede istituzionale della Conferenza unificata Stato-Regioni,

Ora, siamo di fronte ad un ordine del giorno che ripropone il tema del pieno coinvolgimento nel processo decisionale,

che vi sia un atteggiamento di chiusura, che dà anche la cifra del rapporto istituzionale tra Stato centrale e comunità locali su un tema - ripeto ed insisto

contrastato non in maniera ideologica o pregiudiziale ma in maniera assolutamente motivata. Infine, signor Presidente, signor Vice Ministro,

- ci chiediamo come mai questo tipo di investimento - richiamo i colleghi della Lega ad una testimonianza di coerenza - viene poi contraddetto su un tema così importante, su cui le comunità locali non possono che essere coinvolte pienamente. Sulla base di queste motivazioni dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo ordine del giorno e chiedo al relatore ed al Vice ministro

Prego

oscurità delle reali motivazioni che hanno portato il Governo e la maggioranza a decidere il commissariamento della Sogin non mi soffermo, perché già altri colleghi del mio Gruppo al Senato e colleghi deputati del Gruppo PD alla Camera hanno argomentato largamente su questo tema. Mi limito a a descrivere brevemente il contenuto di questi due primi emendamenti, che hanno l'obiettivo, se non altro, di preservare l'operatività della Sogin fino a quando non saranno perfezionate le procedure di rinnovo di rinnovo degli organismi statutari, in un caso mantenendo in carica il consiglio di amministrazione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 7; nell'altro caso, in via subordinata, evitando la cessazione del consiglio di amministrazione di Sogin all'entrata in vigore della legge, posticipandola invece all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Poiché nessuno finora ha capito,

il ruolo e la funzione importante e delicata che svolge ad un pericoloso periodo di interregno, in cui non ci sarebbe responsabilità reale da parte di questa società per azioni. Il terzo emendamento che illustro rapidamente, il 27.6, chiede la soppressione dal comma 47 dell'articolo 27. Il comma 47 è un comma aggiunto nel corso della lettura alla Camera, che presenta contenuti molto gravi perché sostanzialmente depotenzia il ruolo

un soggetto totalmente subordinato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di fatto, come unica facoltà, avrebbe quella di proporre iniziative fase in cui tutto il mondo, a cominciare dal G8 riunito oggi all'Aquila, si interroga sui modi per rendere più spedita, più efficace più utile, anche in termini economici e di innovazione tecnologica, la lotta ai mutamenti climatici, credo che l'aggiunta di questo comma 47 fatta alla Camera sia uno dei tanti segni negativi di questo disegno di legge, che ne fanno un provvedimento in totale ed esplicita controtendenza rispetto alle politiche che in tutta Europa ed in tutto il mondo occidentale si stanno mettendo in campo sul tema dell'innovazione energetica, della lotta ai mutamenti climatici e della cosiddetta *green economy.

tra le *royalties* a terra ed a mare e mettersi contro i Comuni e le Regioni dai quali proviene l'80 per cento del gas, credo sia una logica fuori luogo. Alla Camera un analogo ordine del giorno è stato proposto proposto all'unanimità ed accolto; chiedo pertanto che tale proposta venga accolto anche qui, ma soprattutto chiedo al Governo di rimediare in fretta a qualcosa che è davvero privo di senso.

l'articolo 27 del disegno di legge, in particolare il comma 27, che stabilisce la deroga alle vigenti normative regionali relative alla localizzazione di impianti energetici. questa deroga valga anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione qualora siano allocati in impianti industriali dismessi, nonché per impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva. L'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce poi che per la riconversione a carbone degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di leggi regionali e nazionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, Con questa disposizione, che - si sa - era nata per poter derogare a una norma della Regione Veneto, di fatto si estendono tali deroghe su tutto il territorio nazionale, quindi a tutti gli impianti di carbon fossile di nuova generazione. Vorrei

mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio,

intendiamo ricordare all'Assemblea che è in atto l'estromissione delle Regioni dalle procedure di autorizzazione alla perforazione per la ricerca di idrocarburi.

riteniamo che ciò sia in contrasto con quanto disposto in materia di ambiente, territorio ed energia dalla modifica apportata al Titolo V della Costituzione.

Presidente, vorrei richiamare l'attenzione su un problema che in questi giorni è particolarmente

prorogata la concessione per procedere alle perforazioni di studio e di prova per la ricerca di petrolio e metano. I Comuni si sono pronunciati con grande attenzione, spessore e conoscenza del problema, ma nessuno li ha ascoltati; il disegno di legge esclude gli enti locali, ma il Governo ha appena accolto un ordine del giorno sul medesimo problema e riferito alla stessa zona in cui in sostanza afferma che ascolterà gli enti locali. da me presentato dettaglia dunque una situazione particolare e grave che si sta verificando in uno dei più bei polmoni naturali della Lombardia, in particolare della Brianza. Brianza. Spero che il Governo voglia accogliere anche quest'ordine del giorno, perché sarebbe un segno di chiara attenzione e di interesse verso i Comuni interessati,

e per preservare un'area situata all'interno di una delle zone più urbanizzate e antropizzate d'Italia. la Comunità europea ha ritenuto di identificare questo sito come di interesse comunitario parte di questa zona come parco naturale, mi chiedo come sia possibile che questa stessa area venga assoggettata ad una procedura che renderà possibile una trivellazione per verificare se vi sono idrocarburi.

le zone identificate a tale scopo sono molte, ma distanti da quella individuata. Mi chiedo quindi come sia possibile che una piccola isola, nel cuore della Lombardia, possa essere così importante per una società australiana che si occupa di idrocarburi, quando questa zona è isolata dal contesto che la circonda e soprattutto da quelle aree che invece tradizionalmente in Lombardia vengono considerate

Curone: si tratta di vedere ora se tutti gli interventi che sono stati fatti sulla stampa locale, anche da autorevoli rappresentanti del Governo, trovano davvero riscontro o se invece quello che si dice ai giornali è frutto di parole destinate a perdersi poi nel vento, per cui quello che si fa in quest'Aula o quello che fa il Governo è molto diverso dalle promesse fatte sui territori,

un'indicazione che veniva in maniera unitaria dalla Camera. Mi pare che questo sia un modo di procedere del tutto incomprensibile. Certo è che le Regioni e gli enti locali che si troveranno di fronte a un provvedimento del genere, non staranno in

intervengo per motivare il nostro voto a favore dell'ordine del giorno G27.101, ed anche per segnalare la meraviglia e, in qualche misura, lo sconcerto per la posizione assunta dal relatore e dal Governo. Stiamo producendo atti e dichiarazioni con le quali annunciamo l'obiettivo di potenziare le politiche per l'efficienza energetica, per il risparmio e per la produzione da fonti rinnovabili. Accade spesso che vengano mobilitate ingenti risorse finanziarie per sostenere tali sforzi e per incentivare attività ed impianti di questa natura. In questo caso, si chiede semplicemente di organizzare l'impianto normativo perché possa essere riconosciuta, alla pari delle reti di utenza per gli utilizzatori industriali, la comunità di utenti costituita dai soci delle cooperative non solo di proprietà delle abitazioni, ma dei soci di quelle forme giuridiche

la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree condominiali e in aree gestibili attraverso quelle forme giuridiche, tanto da poter gestire anche lo scambio sul posto dell'energia prodotta e dell'energia consumata, quindi senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Organizzare un impianto normativo che abbia quella finalità

«La notizia secondo cui il Ministero delle attività produttive avrebbe consentito ad un'azienda australiana di effettuare perforazioni nel Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone è ancora da verificare e in questo senso intendo chiedere informazioni al ministro Scajola. Scajola. Nel caso in cui questa notizia venisse confermata» - e lo è - «va da sé che tutta la Lega sarebbe fortissimamente contraria. Il Parco del Curone è un ambiente incontaminato, all'interno del quale gli abitanti non sono nemmeno liberi di scegliere le piante per il giardino della propria abitazione, perché soggetti alle scelte del Parco. È chiaro che queste trivellazioni sarebbero del tutto incompatibili con la bellezza del paesaggio». Allora, la dichiarazione è del senatore Castelli, che mi risulta ancora componente autorevole di questo Governo, se non è intervenuto qualche qualche cambiamento. In Commissione, i senatori Bodega e Monti hanno addirittura chiesto di firmare il nostro ordine del giorno. Vorrei sapere

trascrive alla lettera una delibera del Consorzio di gestione del Parco, nel quale siedono i sindaci, non tutti del PD, dei Comuni di Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego, Rovagnate, Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Sirtori e Viganò. Mi dovete spiegare com'è possibile che in quelle zone si continui a dire che qualcuno vince

e qui non si abbia neppure il coraggio di accogliere un ordine del giorno che ripete semplicemente un deliberato del Consorzio del Parco, nel quale siedono sindaci del PdL, della Lega e del PD. A questo punto, mi chiedo perché il senatore Castelli abbia dichiarato che tutta la Lega sarebbe fortissimamente contraria all'ipotesi di trivellazione all'interno del parco naturale, non in una zona industriale.

Benissimo, allora, visto che sono stato provocato, voterò contro questo ordine del giorno.

nel testo che fu licenziato dal Senato fu introdotta una specificazione circa la natura dell'Agenzia, che mi pare non debba essere sottovalutata. Nel testo licenziato dal Senato, al comma 3, era scritto: "L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato". continuava dichiarando che l'Agenzia avrebbe svolto quelle funzioni senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica

la maggioranza abbia voluto cancellare questa dichiarazione di indipendenza e di autonomia dell'Agenzia che ha una funzione strategica a tutela degli interessi nazionali, della salute dei cittadini e della salvaguardia della qualità ambientale. Per questo motivo noi proponiamo di ripristinare tale dichiarazione di indipendenza e di autonomia dell'Agenzia, proprio perché la materia nucleare richiede le massime garanzie di trasparenza e di certezza che solo un'Agenzia qualificata ed indipendente, alla pari delle Autorità costituite nel nostro Paese, può garantire all'opinione pubblica, ai cittadini, ai portatori di interessi. *(Brusìo)*. [**Presidenza della

perché possa essere ripristinata una norma che, ripeto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

di tranquillità che devono essere garantite attraverso la costituzione e l'operatività dell'Agenzia nucleare, che deve allinearsi ai migliori standard internazionali, osservando i criteri direttivi offerti dall'Agenzia internazionale per l'energia nucleare anche rispetto

e possa adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere più matura la politica e la strumentazione tesa a garantire la sicurezza dei nostri dei nostri cittadini. Vorremmo richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza perché si riconsideri un aspetto fortemente lesivo della credibilità di un'operazione che, già per altre componenti, risulta piuttosto audace, velleitaria e in qualche misura superficiale, come verrebbe confermato dalla contrarietà

L'interrogazione fa riferimento a più eventi calamitosi che si sono verificati nella Regione Basilicata, in questo caso nella Provincia di Matera, nei giorni 2, 4, 18 e 28 maggio 2009, eventi grandinosi che hanno danneggiato le colture in atto in alcuni Comuni. In particolare, la grandinata che si è verificata nel pomeriggio del 28 si è abbattuta su una vasta area della Provincia, interessando anche le colture già colpite da precedenti eventi calamitosi. L'ultimo evento è stato di notevole intensità, con chicchi della grandezza di noci caduti in assenza di acqua e quindi con un elevato potere

i territori interessati ed ha quantificato i danni per il riconoscimento dello stato di calamità, vorrei sollecitare il Governo per sapere se rispetto a questa grave situazione non ritenga opportuno dichiarare con urgenza

intervengo per pregarla di sollecitare il Governo a rispondere a due interrogazioni che ho proposto al ministro della giustizia Alfano,

interrogazioni che chiedono al Governo di rispondere sulla situazione del carcere Dozza di Bologna e delle carceri in Italia in generale. La situazione del carcere della città di Bologna è drammatica. Questa mattina, a Bologna, si sono riuniti in manifestazione tutti i sindacati di polizia penitenziaria e si è svolta una manifestazione nazionale per lamentare la gravissima carenza di organico della polizia penitenziaria, che colpisce tutte le carceri a livello nazionale. Gli organici sono ridotti a poco più della metà di quelli previsti dalle piante organiche. Le condizioni delle carceri in Italia rispetto al problema del sovraffollamento sono drammatiche: oltre la metà degli istituti penitenziari italiani vede una presenza superiore del 40-50 per cento rispetto alla propria capienza, e

il Governo a riferire sulla situazione drammatica che si è venuta a determinare nel mondo della cultura e dello spettacolo dopo l'incauta promessa di inserire nell'ultimo decreto, per così dire, anticrisi, un fondo parzialmente restitutivo dei tagli veementi che un anno fa furono apportati al Fondo unico per lo spettacolo dal cosiddetto decreto Tremonti.

il film italiano, tanto decantato, è ormai ridotto a poco. Il ministro Bondi, che in un più di una circostanza si era dichiarato interessato e anzi favorevole a fare con tutti come si dice in gergo, in modo *bipartisan* - una battaglia per ripristinare il FUS (Fondo unico per lo spettacolo), si è poi reso "latitante". Egli venga a dirci come mai, dopo che il suo Governo non ha fatto quello che era stato promesso,